La seduta e` ripresa.

Presidente, vorrei ricordare che nella scorsa legislatura, nonostante una maggioranza soverchiante di 40 o 50 senatori, molto spesso non si e` svolta la seduta per mancanza del numero legale. credo che non ci sia niente da polemizzare su questa vicenda.